informo la S.V.» – (Brusio) abbassiamo il volume altrimenti ecomplicato – «che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, e stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai rispettivi Sottosegretari di Stato per i medesimi Dicasteri dott. Mario GIRO, on. Teresa BELLANOVA e sen. Riccardo NENCINI.

con l’auspicio, da qui al prossimo 8 marzo, di ricordarci ogni giorno del merito e del valore delle donne. Buon 8 marzo a tutte le senatrici.

testi e letture messe sistematicamente al bando dal sistema intellettual-culturale prevalente in quel periodo. Vorrei ricordare che questo studioso, che e andato sempre controcorrente e che si edistinto per il coraggio delle idee che ha professato,

ubicato in Svizzera che accoglie tutti i premi Nobel per l’economia, soprattutto quelli che vengono dalla scuola liberale.

che rivendicava la supremazia della visione marxista e statalista dell’economia e dello Stato. Oggi e semplice definirsi liberale, ma dobbiamo a gente come il professore Ricossa e all’istituto «Bruno Leoni» la possibilita` di comprendere i guasti delle teorie keynesiane, dello Stato massimo, dell’uso dissennato della leva della spesa e del debito pubblico, che oggi stiamo pagando con la crisi economica. Ritenevo giusto onorare in questa Assemblea questo uomo di scienza, questo pensatore corposo, che ha sempre rifiutato cariche politiche, ma che merita il rispetto e la considerazione di chiunque ama, qui e fuori di qui, definirsi liberale. (Applausi

non necessariamente in contrapposizione al filone keynesiano, egualmente liberale – va ricordato come un grande animatore del dibattito politico, sulle colonne della Stampa, all’universitae

dalla Camera dei deputati, di cui ha fatto parte per due legislature. Vorrei ricordarlo brevissimamente, in questa sede, per il ruolo che ha avuto, limitandomi ad un solo aspetto della sua multiforme e operosissima

proprio in questo ramo del Parlamento la loro parte piu impegnativa nella scorsa legislatura. Domenico Maselli estato molto a lungo professore di storia del cristianesimo a Firenze e ha vissuto gran parte della sua vita a Lucca, dove e scomparso lo scorso sabato. PRESIDENTE.

le vorrei assicurare che il Presidente del Senato ha formalmente rappresentato la sua richiesta al Governo, quindi il Presidente e` in attesa di un riscontro e di un esito di questa formale richiesta.

debbo prospettarle la necessita` di un’inversione dell’ordine del giorno, perche´ non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio sulla riformulazione. Ci sono dei pareri sospesi, quindi le chiederei l’inversione dell’ordine del giorno.

ha preso in esame gli emendamenti registrando un parere positivo del rappresentante del Ministero dell’economia presente in Commissione, senza tuttavia il supporto di una relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria che – ci hanno assicurato dal Ministero dell’economia – ci sara` domattina. Pertanto contiamo

mi riaggancio a quanto ha dichiarato il senatore Caliendo per dire che effettivamente non ci estata data la possibilita

di 56,81 euro per ogni richiesta di rinvio a giudizio; e, invece, prevista una indennita di 10 euro per il provvedimento di archiviazione. Ora, io non voglio mettere in discussione la onorabilitadei giudici di pace, pero se un giudice di pace emette un provvedimento di rinvio a giudizio incamera circa 56 euro; se emette un provvedimento di archiviazione incassa 10 euro. Qualche diffidenza

comunque, con propri emendamenti, cercare di evitare che i cittadini vengano rinviati a giudizio per la soddisfazione di interessi economici di taluni.

signora Presidente, questo provvedimento, che mi sembra abbia trovato una discussione proficua tra le parti politiche, forse, oltre che dell’approfondimento, avrebbe bisogno dell’onesta intellettuale, che credo ci sia da parte del relatore. Per quanto il senatore Cucca

in un dialogo, come e stato provato in questi giorni – dovrebbero consentire a tutti di dire che, a parte l’inadempienza del Governo nel presentare la relazione tecnica (che forse non ecosı marginale nel momento in cui si vogliono presentare e portare avanti dei provvedimenti), un’ulteriore un’ulteriore riflessione, non unicamente legata al rinvio tecnico-politico per la mancanza della relazione, non sarebbe una cosa negativa. Sentivo prima l’intervento del collega Falanga: ci sono delle falle che sono forse risolvibili. Mi piacerebbe, Presidente, fare una domanda che mi permetto di porre in maniera indiretta al relatore. Preso atto che ci sono alcuni problemi che possono essere risolti, c’eda parte del relatore, e quindi del Governo, la volonta di recepire le correzioni in fase emendativa? Infatti se manca questa volontadiventa

non ho difficoltaad aderire alla proposta del collega Cucca, fortificata dal Presidente della Commissione bilancio,

il nostro ordine del giorno, fin da quando e stato pensato, aveva previsto che l’informativa sulla Libia

gli allievi e i docenti dell’Istituto comprensivo «Antonio De Curtis» di Aversa, in provincia di Caserta che assistono ai nostri lavori. Benvenuti a tutti.

Io penso che la riflessione sulle missioni possa comportare la necessita di ascoltare prima cosa diciamo sulla Libia. Non mi sembra un fatto cosıassurdo. Quindi, mi permetto di sollevare questa eccezione, non per non andare avanti su un provvedimento, ma perche´ vi e una logica

il tema delle missioni militari. Questo e un problema di ordine generale, che non ha alcuna connessione con fatti specifici. Domani mattina, invece, come richiesto da molte forze politiche, non ultimo da alcuni senatori nell’ambito della mia Commissione, il ministro

autorizzativa alle missioni internazionali che verranno. Siccome si parlera in Parlamento di come autorizzare queste missioni internazionali, e si autorizzeranno anche missioni in Libia, io ritengo sia necessario ascoltare il ministro Gentiloni al riguardo.

Presidente, illustro l’emendamento 2.7, che vuole riportare la centralitadelle decisioni sulle missioni internazionali al Parlamento, e dichiara semplicemente che le Camere possono negare l’autorizzazione alle missioni internazionali. Niente di piu e niente di meno.

In realta`, il voto sarebbe personale.

ci sembra opportuno capire. Visto che, come diceva il presidente Casini, non c’econtinuita tra quello che facciamo oggi e la presenza domani del Ministro

fare chiarezza. Dunque, vi e un emendamento del relatore che estato riformulato; in quanto tale, deve essere riesaminato dalla Commissione bilancio; la riformulazione e stata mandata ai Gruppi, che

Signora Presidente, le regole vanno applicate perche´ e` stato proprio il Presidente del Senato a voler rimarcare questa cosa. Quindi, prima di procedere

(meglio conosciuto come IDI), il San Carlo di Nancy e Villa Paola. Al centro dell’inchiesta per fatti illeciti e appropriazioni (avvenute in danno soprattutto dell’IDI tra il 2007 e il 2012) c’el’attivita di padre Franco

tutti furono arrestati nell’aprile 2013. Numerosi sono gli episodi di distrazione dei fondi ai danni della Congregazione. L’inchiesta prese le mosse da un esposto nel quale alcuni dipendenti dell’IDI lamentavano il mancato versamento degli stipendi e segnalavano una serie di incongruenze nella gestione amministrativa. Sul fallimento dell’IDI e del San Carlo di Nancy io stesso ho presentato un’interrogazione ai Ministri della salute e dello sviluppo economico ho partecipato ad alcuni degli innumerevoli presidi dei lavoratori, che ancora una volta risultano essere la parte piugravemente lesa da sciagurate operazioni fallimentari e patrimoniali. Si e prospettata persino la possibilitache proprio i soggetti responsabili del fallimento delle suddette strutture potessero ricomprare, tramite la fondazione Luigi Maria Monti, costituita

Non e possibile che a pagare il prezzo di corruzione e malaffare siano ancora una volta i lavoratori e le loro famiglie. Il tessuto vivo della citta, in un momento di recessione e stagnazione, si ricostruisce anche puntando sulla ricerca e sulle eccellenze mediche. Ma, per farlo, e necessario restituire rispetto, valore e dignitaal prezioso lavoro di tante persone che in questi mesi durissimi non si sono arrese e hanno continuato, a volte solo sulle proprie forze, il lavoro di cura e accoglienza sul territorio. Infine, leggo che la Regione Lazio si costituira parte civile, e questo eun bene. Chiedo che il Ministero e la Regione Lazio si assumano la responsabilita, coinvolgendo innanzitutto le organizzazioni sindacali – esse esse rappresentano le donne e gli uomini che, negli ultimi anni, spesso da soli, hanno tenuto in vita questi importanti presidi – di individuare un percorso che difenda e rilanci, con il contributo del Vaticano, realtache in pieno Giubileo della Misericordia tenete conto che esse si trovano a poche centinaia di metri dalla Basilica di San Pietro – rappresentano i primi poli di riferimento per milioni di cittadini italiani e pellegrini di tutto il mondo. Occorre farlo ora, adesso, perche´ non c’e piu` tempo da perdere.

una mozione per chiedere al Governo di procedere agli opportuni controlli preliminari allo scioglimento del Comune di Maddaloni, in provincia di Caserta, per fatti che noi riteniamo gravissimi e che voglio qui far presente. Ieri estato arrestato il sindaco di Maddaloni Rosa De Lucia, assieme ad un assessore, due consiglieri comunali un imprenditore nel settore dei rifiuti. Come comunicato dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, il sindaco utilizzava l’imprenditore Di Nardi come un vero e proprio bancomat, dal quale incassava tangenti anche a suo piacimento, ovvero dietro le sue stesse richieste. Queste tangenti venivano poi utilizzate dal sindaco per comprare il consenso dei consiglieri comunali, ottenendo l’approvazione del bilancio e altri fondamentali atti amministrativi che, se non approvati, avrebbero causato lo scioglimento automatico del Comune. Il sindaco si assicurava, dunque, la maggioranza per restare in carica e il consenso dei consiglieri comunali, mediante pratiche corruttive organizzate a tal punto che ogni consigliere aveva il suo prezzo di acquisto, venivano somministrati nella misura del 50 per cento prima del voto e il restante 50 per cento a votazione avvenuta. Inoltre, come spiega la procura, il sindaco conduceva la macchina amministrativa anche comprando il consenso degli imprenditori locali, affidando loro, in modo diretto e in prima persona, servizi e forniture di eventi organizzati nel Comune, senza alcuna regola, per risultare ben vista agli occhi dei suoi concittadini e ottenere evidentemente la sua rielezione a sindaco. Infine, piegava alla sua volonta i funzionari comunali rimuovendoli dai loro uffici e costringendoli dunque ad eseguire modifiche agli atti amministrativi, come nel caso dell’annullamento delle penali, inflitte dal funzionario responsabile del servizio ambiente ed ecologia del Comune, contro la ditta DHI, che poi corrispondeva appunto le tangenti al sindaco attraverso il suo titolare Di Nardi. Signora Presidente, emerge dunque una tangentopoli locale che parte dall’interno del Comune e coinvolge anche all’esterno tutti gli strati sociali, di cui la stampa locale narra anche quotidianamente sulle sue pagine, a riprova che il malcostume e la corruzione sono cosa risaputa da tutti. La procura scrive che alcuni consiglieri comunali, oggetto delle tangenti elargite, non sarebbero ancora stati individuati. individuati. Per tutti questi fatti esposti ed accertati dalla magistratura auspichiamo che venga al piupresto ripristinata la legalita, attraverso lo scioglimento immediato del Consiglio comunale del Comune di Maddaloni. Signora Presidente, gentili colleghi, desidero sottoporre all’attenzione di quest’Assemblea la delicata situazione relativa al litorale della costa adriatica Il Pilone, 8 marzo 2016 E[]doverosa una premessa: il Comune in oggetto, Ostuni, e considerato una delle perle del Mediterraneo, per le bellezze paesaggistiche e ambientali del territorio. Per queste caratteristiche, euno dei punti di maggior richiamo turistico della costa adriatica e del Salento. A minacciare la bellezza della spiaggia di Torre San Leonardo-Il Pilone sarebbe il progetto dell’Acquedotto pugliese, un progetto che prevede l’adduzione di una fogna proprio nella localita costiera. Sı, gentili colleghi, si tratta dell’ubicazione di una vasca in cemento armato di raccolta e delle pompe di sollevamento dei reflui letteralmente a ridosso della spiaggia del Pilone. La vasca di liquami incriminata prevede, di fatto, la canalizzazione fognaria della costa nord di Ostuni. Questo scempio rischia di compiersi, se non si interviene immediatamente. Sono valse a poco le mobilitazioni dei cittadini, le denunce della stampa, il ricorso al TAR e successivamente al Consiglio di Stato (di cui ancora si attende la decisione) la decisione) e la visita del sottosegretario Degani. Come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, abbiamo gia richiesto un’audizione urgente dei vertici dell’Acquedotto pugliese, dell’Autorita` idrica

Daremo battaglia affinche´ un territorio unico, come quello della costa salentina, meta internazionale di turismo, non venga profanato e mortificato in questo modo.

La sera del 25 febbraio 1992, l’esercito armeno aprı il fuoco sulla cittadina di Khojaly, che rappresentava un obiettivo fondamentale nella strategia di occupazione della regione. In poco meno di un giorno, le precarie difese della cittadina vennero meno. Si organizzocosı un corridoio umanitario per far evacuare i civili. Ma donne, bambini ed anziani, in violazione di fondamentali norme internazionali, vennero uccisi mentre tentavano disperati la fuga attraverso quel corridoio umanitario.

che invocavano il ritiro delle forze di occupazione dalle aree occupate appartenenti alla Repubblica dell’Azerbaijan, nonche´ gli inviti del Parlamento europeo e della NATO a rispettarne il contenuto: contenuto: tutti tentativi che, per ora, non hanno avuto alcun esito e alcuna attuazione. Allo stesso tempo, troppo debole el’attenzione della comunita internazionale verso una situazione che potrebbe degenerare nel breve periodo. Sarebbe dunque importante, e quindi auspicabile, che il Governo italiano nelle sedi opportune riaffermasse l’importanza di iniziative per la soluzione del conflitto del Nagorno Karabakh, ribadendo che il rispetto delle risoluzioni dell’ONU prima citate rappresenta un passaggio fondamentale per proseguire sulla strada di una soluzione pacifica.

2012, che ha sancito la doppia preferenza di genere, nonche´ la legge Delrio, la n. 56 del 2014, che sancisce finalmente l’equilibrio di genere nella composizione delle Giunte. Abbiamo inoltre una legge elettorale europea con la preferenza alternata di genere, e cosı via.

e il nostro pensiero vogliono andare non tanto e non solo alle grandi Costituenti e ai grandi passi in avanti fatti anche in tempi piu recenti nel nostro Paese, grazie all’impegno di tante donne – un Paese senza memoria eun Paese senza storia, senza anima a tutte le donne del silenzio; a quelle donne che, senza clamori, hanno consolidato e trasmesso i valori della solidarieta, dell’amicizia, della famiglia, dell’accoglienza e della dedizione. A loro vanno il nostro pensiero e il nostro alle donne della sensibilita sociale, della dedizione gratuita: quelle belle dentro. E non dimentichiamo le donne del silenzio, le migranti di ieri e quelle di oggi; quelle avvolte da una coperta sotto la pioggia, che cercano una via di fuga dalla guerra e sperano in un’Europa solidale; quelle donne che le immagini veloci di una telecamera distratta sfiorano appena,

si aprano; donne migranti, alla cui condizione va restituita dignita, persone in qualche modo sacre; quelle dell’esodo inarrestabile, che aspettano una risposta politica e umanitaria al confine tra Grecia e Macedonia, davanti a focolari improvvisati in attesa di un improbabile pullman. E[ ]in questo giorno che l’Europa solidale deve affermarsi e prevalere sull’Europa degli egoismi, un’Europa piuattenta al femminile, capace di agire subito piu che di negoziare davanti a un’emergenza senza precedenti.

La seduta e` tolta